è inutile che continuiate a programmare i lavori d'Assemblea senza tenere conto dei lavori delle Commissioni, in particolare della Commissione bilancio (e poi *a posteriori* dire che è colpa della Commissione bilancio se i lavori vengono rallentati). Le Commissioni non possono lavorare

calendario dell'Assemblea senza tener conto della tempistica dei lavori della Commissione bilancio. È ovvio che non riusciamo a stare dietro a tutto.

avrebbe confidato il proprio sì alle riforme costituzionali. Io ho atteso qualche giorno per sottoporre il quesito al Presidente del Senato,

punto 3) il parere è favorevole con una riformulazione: va eliminato il riferimento al decreto direttoriale.

oltre all'illustrazione delle mozioni, compresa quella puntuale e competente che ha fatto il collega Orellana, induce a fare due riflessioni. La prima riflessione vi è un problema di grave criticità all'interno dei percorsi che garantiscono la continuità assistenziale sul versante della garanzia garanzia della somministrazione dei farmaci nelle scuole. È un problema che con sfumature differenti, finanche quelle che con toni precisi e puntuali dell'attualità ha presentato la collega Emilia De Biasi con tono appassionato, dimostra che in effetti c'è un grave *vulnus* e che la continuità assistenziale nella scuola non trova adeguati livelli di risposta, di garanzia e di appropriatezza per una domanda elementare e basilare che lì si rappresenta con riferimento ad una platea di soggetti, proprio i bambini, che sono affetti, come emerso dal comitato paritetico, in particolare da tre patologie: dal diabete, dall'asma e dall'epilessia. È un problema che va risolto. La seconda riflessione è che non ho sentito voci dissonanti in merito alla valutazione delle varie circostanze, al racconto, se mi si consente, che è stato fatto da tutti i colleghi intervenuti - e ringrazio anche coloro i quali hanno espresso il proprio consenso sottoscrivendo la mia mozione nel rappresentare con sfumature differenti l'esistenza del problema. Vi è quindi un problema e vi è l'unanime volontà, signor Sottosegretario, da parte di quest'Assemblea, di porvi rimedio e di farlo con delle richieste che vengono affrontate. Ho accettato la riformulazione che lei, Sottosegretario, ha chiesto; credo che sia di natura meramente formale

deve affrontare con riferimento alla necessità di garantire l'accesso ai presidi inseriti nell'ambito dei *medical device* che consentono un più rapido ed efficace accertamento

si è creato e la frattura che si è evidenziata anche nel dibattito dell'Assemblea con gli articoli 32, 33 e 34 della Costituzione, proprio perché il diritto alla salute deve necessariamente trovare una migliore e più efficace declinazione dei principi costituzionali con riferimento al diritto alla formazione e allo studio. Credo che con questi presupposti il dibattito abbia oggi consentito di consegnare, con il voto favorevole che ci sarà, un impegno che il Governo assume e che è destinato a consentire il conseguimento degli auspicati risultati che saranno risolutivi delle criticità evidenziate. Ciò a beneficio della nostra sanità, ma soprattutto dei diritti della persona, dei bambini e delle loro famiglie che recuperano una condizione di fiducia nelle istituzioni e anche di certezza nel fatto che un bambino a scuola non sia mai in una condizione di abbandono, ma trovi anche nel personale scolastico - attraverso quella generosa vocazione al servizio che noi nella scuola abbiamo sempre considerato fondamentale e che apprezziamo come gesto di vicinanza e di disponibilità del corpo docente e non solo - un presupposto fondamentale per conseguire i risultati che noi tutti abbiamo individuato come necessari per dare una risposta definitiva al problema. Con questi presupposti annuncio il voto favorevole del Gruppo Conservatori e Riformisti alle due mozioni.

Ci rendiamo conto delle difficoltà: stiamo dicendo che dobbiamo formare il personale docente (e non) a fare gli infermieri e i medici. Mi metto nei loro panni quando dovranno iniettare dell'insulina; mi auguro e prego il Signore che non sbaglino il dosaggio: tra «unità» e «cc» basta sbagliare un'unità di misura che bisogna dargli anche l'immunità contro l'accusa di danno, se non di peggio. La questione è molto seria, forse rientra piuttosto nella medicina scolastica. Forse è più opportuno che siano medici e infermieri Grazie,

il costo. Siamo in pediatria: abbiamo un'AIFA con costi del farmaco più alti d'Europa e i familiari non riescono a curare i loro figli per mancanza di risorse.

avanzate anche giuste obiezioni,

Deve sicuramente rimanere la volontarietà da parte dei docenti di assumersi un carico di responsabilità non ordinaria, che non gli compete, ma la cosa è assolutamente fattibile. Potrebbe anche esserci un ausilio di personale idoneo, specifico per questo tipo di

uno scambiarci opinioni e manifestare grandi e importanti principi che però alla fine resteranno sulla carta. Speriamo che, alla fine di questo dibattito, la questione venga definita e concretizzata. la discussione svolta ieri ci ha permesso di approfondire in modo importante la problematica riguardante il diritto allo studio e la salute di ragazzi e bambini affetti da patologie croniche. Si tratta di un argomento molto delicato e difficile. Nella mia esperienza di diabetologo e medico di famiglia ho perfettamente chiaro cosa vuol dire gestire ragazzini e bambini diabetici, in particolare durante le ore di lezione.

indicati nelle mozioni come meritevoli di indicazioni al Governo per essere attuate. difficile quando si parla di microinfusori, che non sono facilmente gestibili e hanno un costo importante, o quando si parla di personale sanitario nelle scuole, di infermieri e di medici, che Grazie, io sono il più contento perché dovremmo poi impiegarli soprattutto per fare prevenzione ed educazione sanitaria a tutti i ragazzi e non solo a quelli più sfortunati.

da patologie croniche (in maniera particolare, in questo caso, da diabete). Proprio perché si tratta di conciliare diritto alla salute e diritto allo studio ci sarebbe piaciuto vedere in quest'Aula, oltre alla sottosegretaria D'Onghia, che ringraziamo,

quante risorse il sistema sanitario nazionale investe nella sanità territoriale, perché non si tratta di aprire dei presidi medici all'interno delle scuole, bensì di garantire, ad esempio, la figura dell'infermiere del territorio che garantisce il diritto allo studio e studio e alla salute nelle scuole. Quindi il punto è quante risorse vengono dedicate dallo Stato alla alla sanità nazionale e soprattutto alla sanità deospedalizzata e quindi al territorio che in questi anni, in seguito ai tagli e alle scelte del Sistema sanitario nazionale e delle Regioni, purtroppo è stato fortemente penalizzato e continuerà ad esserlo

Grazie,

Presidente, ieri, nel corso della discussione generale sulle mozioni, tra le varie criticità che sono emerse abbiamo riscontrata una che, secondo noi, merita anche oggi una piccola precisazione ed è quella relativa al fatto che sia nelle scuole elementari che nelle scuole medie molte volte vengono richiesti interventi d'urgenza,

Vede, signor Sottosegretario, questa patologia, come già abbiamo avuto modo di sottolineare quando abbiamo discusso sull'obesità, secondo noi anche in questo provvedimento meriterebbe particolare attenzione per il semplice fatto che ormai è noto a tutti, non solo per le direttive dell'Organizzazione mondiale della sanità ma anche per le direttive delle organizzazioni medico-scientifiche, da l'obesità infantile costituisce un quadro prodromico importante, pericolosissimo per quanto riguarda l'obesità in età adulta e quindi con costi enormi per il Sistema sanitario nazionale. riteniamo che gli interventi di prevenzione siano importanti, soprattutto nel caso di specie, e che debbano partire dalla riorganizzazione e dalla rimodulazione del sistema della prevenzione, soprattutto nelle scuole. ancora una volta l'esperienza passata che introduceva nei dipartimenti di prevenzione le unità operative di educazione sanitaria e soprattutto di medicina scolastica

proprio in virtù del fatto che molte risorse potrebbero essere risparmiate e reinvestite per migliorare l'organizzazione del sistema sanitario ma anche la riorganizzazione dei rapporti tra sistema scolastico e sistema sanitario. *(Applausi dal Gruppo* *AP (NCD-UDC) e del senatore Di

sono rimasto abbastanza sorpreso e preoccupato dalla discussione che si è svolta nella giornata di ieri e, soprattutto, sono preoccupato e sorpreso

si fanno merito degli onori quando devono andare a tagliare i nastri e cioè raccogliere gli applausi e, al contrario, scappano quando ci devono mettere la faccia. Questo è uno degli esempi.

modificazioni notevoli), venne istituito un Comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci a scuola;

e, soprattutto, all'impegno delle famiglie, i cui membri spesso per assicurare questo tipo di trattamento devono prendere lunghi periodi di aspettativa e, in alcuni casi, lasciare il posto di lavoro. Dunque, lo Stato deve farsi carico di tutto questo. non si capisce però perché, nel 2016, malgrado questo Comitato paritetico abbia concluso i propri lavori e malgrado le associazioni di categoria, sia delle famiglie che del corpo scolastico, abbiano sollecitato l'approvazione di queste linee guida, il Governo non abbia ancora approvato e fatto pubblicare le linee guida fondamentali, lasciando ancora una volta le famiglie e il personale a dover rispondere a queste esigenze. Ha ragione la senatrice

Non ci si può fare sempre portavoce della difesa del sistema sanitario nazionale, dell'universalità del sistema sanitario nazionale, per cui nessuno viene lasciato solo,

Per queste motivazioni, il voto di Forza Italia sarà favorevole ad entrambe le mozioni perché, almeno, hanno manifestato la volontà di un superamento delle difficoltà, cosa che il Governo non fa. sono state presentate e discusse due mozioni che prendono lo spunto da uno stesso problema: entrambe pongono all'attenzione un grande problema che si trascina da anni, che molte Regioni hanno saputo risolvere da tempo, con ottimi risultati, ma per il quale in altre Regioni ancora tutto è lasciato indefinito. Si tratta dell'inserimento a scuola del bambino con il diabete di tipo 1 e della relativa gestione durante l'orario scolastico, problema che tocca aspetti come la somministrazione del farmaco indispensabile (ovvero l'insulina) e la somministrazione al bisogno del farmaco salvavita (il glucagone): evento, quest'ultimo, che in realtà si verifica molto raramente, in particolare durante l'orario scolastico. Non dimentichiamo poi che tale questione tocca anche aspetti psicologici, quelli propri di una patologia come il diabete di tipo 1 che, tipicamente, non si vede, se non nel momento della misurazione della glicemia e nella somministrazione dell'insulina. Si tratta di un problema, dunque, che non si esaurisce individuando *tout court* chi debba somministrare un farmaco, ma che richiede l'elaborazione

Si tratta di un problema che interessa tanti bambini e quindi di un problema che interessa a monte anche le loro famiglie, già provate da una diagnosi di esordio di diabete che all'inizio porta a nascondere il proprio figlio dietro ad un muro di numeri (quelli delle misurazioni della glicemia e delle dosi di insulina), che non ti fa dormire la notte anche per pensare a come poter gestire il figlio anche durante l'affidamento alla scuola, districandosi con il lavoro, per chi ha la fortuna ancora di averne uno. Il ruolo della scuola è fondamentale per consegnare alla

se, mentre gli altri mangiano, ridono e scherzano, lui, dopo magari avere atteso sulla porta della scuola che si materializzasse all'orizzonte l'auto medica, vincitrice degli ingorghi dell'ora di punta, debba poi sedersi a tavola accanto ad un infermiere con la bilancina pesa-alimenti. Cosa gli resta di quel pasto al bambino? Il sistema

per aver recepito le istanze contenute nelle due mozioni, che noi voteremo convintamente a seguito delle riformulazioni proposte dal Governo. Credo davvero che sia importante, per i motivi già esposti esposti da tanti colleghi molto compiutamente, perché credo che non possiamo attendere un minuto di più. Le famiglie ce lo chiedono, le famiglie lo attendono e i bambini ne hanno assolutamente diritto. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione. Passiamo alla votazione della mozione n. 555

l'università, per incentivare i dipartimenti di geologia che spesso hanno pochi professori e anche pochi iscritti. In un momento come questo, in cui, come tutti sappiamo, vi è la necessità di favorire la ricerca nel campo della geologia e di avere più persone e professionisti che si occupano di tale ambito, con questo provvedimento noi incentiviamo i ragazzi ad iscriversi a quelle facoltà nello stesso tempo, semplifichiamo alcuni percorsi all'interno degli atenei in modo tale che si possano costituire dei dipartimenti anche con un numero di professori inferiore rispetto a quello richiesto per tutti

di predisporre un provvedimento che, a questo punto, riteniamo possa essere di sufficiente soddisfazione rispetto alle finalità che si proponeva. Esso è breve. Si compone di tre articoli ed intende sostenere la formazione e la ricerca nel campo delle scienze geologiche e, più in generale, delle scienze della terra. Il testo promuove gli studi in materia di scienze geologiche attraverso incentivi per i nuovi iscritti (anche questo è stato introdotto),

Il miglioramento dell'ambiente e la messa in sicurezza del territorio sono stati inseriti tra gli obiettivi dell'agenda possibile del gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed europea istituito dal Presidente della Repubblica nel 2013. Nel corso dell'esame nella nostra Commissione, sono stati compiuti approfondimenti sulle proposte emendative e sulla copertura finanziaria prevista dal provvedimento, su cui sussistevano alcuni problemi posti dalla Ragioneria generale dello Stato; da qui anche i tempi un po' più lunghi - lo voglio dire qui in Aula - per riuscire a trovare comunque le coperture. Questi emendamenti sono stati approvati in sede di Commissione e ulteriori emendamenti sono stati presentati in sede di Commissione bilancio; quindi diciamo che oggi siamo in grado di esaminarlo in Aula. Nello specifico, al fine di incentivare l'iscrizione di studenti capaci e meritevoli ai corsi di laurea appartenenti alla classe e L34 (scienze geologiche) e ai corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM79 (scienze geofisiche), l'articolo 1 («Incentivi per l'iscrizione a specifici corsi di studio»), in seguito alle modifiche apportate in Commissione, prevede che venga destinata una quota almeno pari a 150.000 euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, nonché del contributo statale erogato alle università non statali legalmente riconosciute, per l'anno 2017. Tali incentivi sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012. L'articolo 2 riguarda «Risorse per progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica» intende sostenere - come dicevo prima - la ricerca per la previsione e prevenzione del rischio idrogeologico, con due diverse tipologie di finanziamento. Per quanto concerne la prima tipologia, si parla di una percentuale del fondo per la prevenzione del rischio sismico che è riservata al finanziamento dell'acquisto, da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati ogni anno dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. che tale fondo risulta istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che quindi questi fondi possono presumibilmente essere messi a disposizione anche per il futuro. La seconda tipologia di finanziamento consiste in un'autorizzazione di spesa di un milione di euro per l'anno 2016. Qui ci sarà una modifica, perché la previsione di spesa era per l'anno 2016

che per la costituzione di un dipartimento universitario è necessario un numero minimo di 35 unità tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, che viene elevato a 40 nel caso di atenei con oltre 1.000 professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei. Con al nostro esame disponiamo che si possano costituire dipartimenti universitari con la presenza anche di soli 20 professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato (quindi, non più di

Questo articolo, come comprendete bene, colleghi, è finalizzato a consentire la costituzione di dipartimenti universitari anche nel caso in cui afferisca ad essi un numero minore di docenti e ricercatori. Questa è stata la richiesta e abbiamo considerato di voler attuare questa disposizione proprio perché i dipartimenti di scienza della terra da molti anni

ha determinato una notevole contrazione del numero di dipartimenti di scienze della terra nei vari atenei d'Italia (esattamente il contrario di quello che servirebbe al nostro Paese) e quindi il conseguente accorpamento con altre discipline non appartenenti alla medesima area disciplinare. Vogliamo, invece, dare nuovamente un'identità forte a questo settore disciplinare, proprio per le necessità che abbiamo nel nostro Paese, così esposto a rischi di varia natura (idrogeologici, sismici e

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

meritano l'attenzione dell'Assemblea, non fosse altro per la cogente necessità di provvedere a dotare il Paese di ulteriori intelligenze, capacità e competenze nello studio delle scienze della terra e, particolarmente, della geologia. Provvedere, però, con un apposito provvedimento *ad hoc* alla incentivazione degli studi geologici, quindi anche delle professioni della della scienza della terra, significa anche denunciare all'opinione pubblica e al sistema Paese (dal punto di vista di chi ha l'obbligo, se non la responsabilità, di provvedervi)

In questo provvedimento si incide su due fondi. Il primo è il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e il secondo è il Fondo per la prevenzione del rischio sismico. Sul primo si incide

cinquant'anni dalla tragica alluvione di Firenze e della Toscana e anche del Veneto e di Venezia, che

preservazione dei beni culturali e dell'integrità fisica e morale del Paese servono geologi ed esperti nel settore delle scienze della terra. Io avrei previsto ulteriori fondi

al reclutamento. Sono pochi e andrebbero aumentati in quanto una seria azione di reclutamento prevede

ha nuovamente riportato al centro dell'attenzione generale la fragilità del territorio italiano e la sua elevata esposizione ai rischi geologici. Periodicamente gli eventi naturali che funestano con regolare puntualità il nostro Paese riportano alla ribalta l'importanza del ruolo del geologo. È triste pensare che ci si ricordi di questa figura professionale e scientifica sempre a disastro avvenuto, nel momento della conta delle vittime e della valutazione dei danni materiali alle attività economiche, agli edifici ed alle infrastrutture. Nella certezza che finalmente si sia raggiunto un punto di svolta culturale - e di questo è testimone l'impegno profuso dal Governo con il varo del progetto Casa Italia - va ricordato quanto sia importante la prevenzione nella mitigazione dei rischi rappresentati da eventi calamitosi di origine geologica. Per attuare una corretta ed efficace attività di prevenzione dai rischi geologici è fondamentale il ruolo della conoscenza del territorio che permette di formare un cittadino consapevole del contesto in cui vive. La capillare presenza di dipartimenti di scienze geologiche distribuiti sul territorio nazionale riveste quindi un ruolo fondamentale per la formazione sia di professionisti geologi esperti in materia sia di insegnanti che possano divulgare la conoscenza geologica nelle scuole di ogni ordine e grado, dove si dovrebbe avviare la formazione consapevole dei cittadini di domani. n. 1892, che ci apprestiamo a votare, una volta divenuto legge dello Stato italiano sicuramente non risolverà di colpo tutte le condizioni di rischio geologico del Paese, ma potrà essere un primo strumento utile per rilanciare il ruolo del geologo a tutti i livelli nella comunità tecnico-scientifica nazionale e per contrastare la forte contrazione che la comunità accademica delle scienze geologiche sta subendo da diversi anni, nella speranza che queste poche risorse e strumenti che stiamo mettendo a disposizione non siano un intervento ormai tardivo.

probabilmente meglio lo sviluppo di alcune discipline che riguardano pochi docenti, proprio perché l'interazione e la prossimità con altre discipline permettono uno sviluppo migliore.

Riteniamo che il disegno di legge in esame giunga opportuno nel recepire le istanze provenienti dal mondo delle professioni del Paese allo scopo di poter incentivare studi, ricerche e professionalità nell'ambito complesso delle scienze della terra. Inoltre,

parte delle intelligenze e dei talenti che insistono nel nostro Paese verso questo tipo di studi.

bene ha fatto la relatrice a prevedere premi e buoni studio per incentivare, fino all'anno scolastico 2020, le iscrizioni alle facoltà di scienze e tecnologie geologiche, scienze geologiche

i danni ad evento avvenuto. Quindi, come in medicina si dice che prevenire è molto meglio che curare, questo disegno di legge stanzia risorse dà le impostazioni legislative per prevenire i disagi e i danni geomorfologici e idrogeologici sul nostro territorio. Correttamente, quindi, anche il nostro Gruppo del senatore Bocchino,

oggigiorno avrebbe il coraggio di opporsi a un provvedimento che prevede qualche spicciolo in più per un settore strategico per il nostro Paese, e cioè quello della prevenzione

per poter disporre di qualche ulteriore spicciolo per i laureati in scienze geologiche. Probabilmente bastava una decisione ministeriale, così come probabilmente non c'era neanche bisogno di una legge per disporre di destinare una piccola parte del Fondo di prevenzione del rischio sismico,

il disegno di legge che stiamo per votare affronta due temi che rispondono alla stessa *ratio*. Il primo tema è favorire e incentivare lo studio delle scienze geologiche, facilitandone l'accesso universitario agli studenti capaci e meritevoli. Si tratta di un settore di studio molto specialistico, apparentemente con non grandi prospettive occupazionali per chi consegue questo tipo di laurea. Su questo, però, è opportuna una riflessione. Gli eventi sismici che hanno interessato l'Italia poche settimane fa, ma anche negli anni scorsi e in tempi più lontani e che periodicamente interessano l'intero globo terrestre, inducono a una riflessione su come sia necessario poter disporre di tecnici adeguatamente formati. Conoscere i processi che determinano l'evoluzione tettonica del nostro Pianeta, i processi di modellamento dei versanti, il ciclo litologico e le dinamiche alla base dei fenomeni sismici e vulcanici significa comprendere i rischi intrinseci al Pianeta. La Terra è un sistema assai complesso, in cui le variabili fisiche, chimiche e biologiche agiscono profondamente sull'ambiente, alterandone in misura spesso significativa i processi evolutivi. Comprendere quali siano i rischi legati alla costruzione in zone sismiche, o in aree ad alto rischio idrogeologico, è utile per prevenire le catastrofi a cui ho appena fatto riferimento. Studiare quindi i processi che plasmano e cambiano la Terra assume grande rilievo se viene visto nell'ottica di poter prevenire i rischi che periodicamente si presentano. La geologia è scienza importante anche per la previsione e la comprensione dei pericoli naturali, per l'individuazione e il risanamento dei problemi ambientali, per la pianificazione territoriale, per la realizzazione di opere pubbliche e private e per lo studio sui mutamenti del clima e dell'ambiente. Molteplici sono quindi i campi di applicazione e favorirne lo studio diventa un investimento per il futuro, sia dell'ambiente che dei singoli territori. disegno di legge è il finanziamento per l'acquisto da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca di strumentazioni tecniche moderne che consentano di approfondire gli studi per la previsione e la prevenzione dei rischi geologici. È un campo, quello dei laboratori e delle strumentazioni nelle scuole, molto delicato, per la precarietà che spesso si incontra, e non solo nelle scuole superiori di indirizzo tecnico, ma anche nelle università. È previsto inoltre il finanziamento di progetti di ricerca presentati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca e questo non può che essere di grande importanza in un momento in cui spesso, e forse troppo spesso, parliamo di cervelli in fuga, a causa della limitatezza dei fondi destinati alla professionalizzazione dei ricercatori e ai progetti di ricerca. Da rilevare, poi, è l'aspetto di carattere normativo,

su cui è stato sollecitata una perplessità da parte del senatore Dalla Zuanna. Condividendone lo spirito, e proprio per evitare che quanto approviamo oggi inneschi un meccanismo di emulazione di tale previsione, credo sia necessario ribadire la specificità e le motivazioni contingenti di tale opportunità. Nonostante la semplicità e la condivisione del disegno di legge - come ricordato anche da parte di altri Gruppi il provvedimento ha avuto un *iter* lungo, se pensiamo che è stato assegnato alla 7a Commissione a maggio dello scorso anno; il parere non favorevole da parte della Ragioneria generale dello Stato ha poi reso necessario modificarne in parte i contenuti.

*(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, questo disegno di legge ha una sua rilevanza, perché vuole sostenere la formazione e la ricerca nel campo delle scienze geologiche, e più in generale delle scienze della Terra, promuovendo queste ultime nel mondo studentesco, anche con il finanziamento per la realizzazione di progetti *ad hoc*. La tutela dell'ambiente e la messa in sicurezza del territorio dovrebbero essere una priorità di qualsiasi Governo, ma negli ultimi anni non è stato così, nonostante l'Italia sia purtroppo un Paese riconosciuto ad alto rischio geologico e idrogeologico, cento della popolazione che vive in zone ad alto rischio sismico e ben 6 milioni in aree pericolose dal punto di vista idrogeologico. Non meno eloquenti e allarmanti risultano i dati pubblicati dall'ISPRA: cento del territorio nazionale è stato interessato da frane. Terremoti e frane causano vittime, feriti e danni a edifici, abitazioni, infrastrutture e beni culturali. Addirittura, nel biennio 2014-2015, oltre i gravi terremoti, si sono verificati più di 200 eventi franosi, per non parlare del rischio idraulico, associato inevitabilmente al verificarsi di frane e smottamenti: ben 12.218 chilometri quadrati di territorio nazionale sono caratterizzati da elevata pericolosità idraulica. Ben venga, quindi, la volontà, presente in questo disegno di legge, di incentivare l'iscrizione di studenti, capaci e meritevoli, ai corsi di laurea in scienze geologiche, scienze e tecnologie geologiche e scienze geofisiche, attraverso la destinazione *ad hoc*, a decorrere dal 2017, di una quota pari a 150.000 euro del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e del contributo statale erogato alle università non statali legalmente riconosciute. Ben venga questo, perché andiamo a valorizzare la meritocrazia. E ben venga anche la destinazione dell'uno per cento del fondo per la prevenzione del rischio sismico al finanziamento dell'acquisto, da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, della

la collega, relatrice Di Giorgi, avrebbe auspicato un maggior impegno, ma il Governo è stato un pochino corto un aspetto questo che, dopo il verificarsi di eventi calamitosi, come quello di Amatrice, è sempre stato considerato prioritario nelle intenzioni, ma è stato poi disatteso nei fatti. Nel disegno di legge in esame c'è un'ulteriore forma di finanziamento per i progetti di ricerca voluti da università ed enti pubblici di ricerca, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, con una spesa di 1 milione di euro per il 2016 (che poi è stato spostato) e di 2 milioni di euro per ciascun anno, fino al 2018. Si tratta di una disposizione importante, così come nell'articolo si consente di porre fine all'accorpamento dei dipartimenti di scienze della Terra con altri dipartimenti non afferenti alla medesima area disciplinare, consentendo di recuperare una specificità che, a causa delle limitazioni imposte dal *turnover* e a quelle previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la costituzione di un dipartimento universitario, era ormai andata perduta. L'articolo 3, infatti, permette la costituzione di dipartimenti universitari di soli venti professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato (e non necessariamente di 35, come stabilito dalla legge n. 240 del 2010), purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento del totale del corpo docenti e ricercatori di quell'indirizzo universitario, consentendo quindi anche la ricostituzione di quei dipartimenti, come scienze della Terra, che erano scomparsi o accorpati ad altri dipartimenti. Condividiamo pienamente, quindi, nel complesso la *ratio* del disegno di legge, anche se abbiamo dovuto evidenziare una mancanza di fondi più incisivi e strutturali. Ad ogni modo, con il nostro Gruppo ci auguriamo che fra tre anni le risorse siano nuovamente stanziate ed esprimiamo voto favorevole. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Guglielmo Marconi» di Terni, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti al Senato e grazie della vostra visita.

nell'attività molto intensa, ma spesso trascurata, di prevenzione, studio e previsione del rischio geologico. Noi stanziamo molti soldi

che è nelle dirette disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze, che peraltro è in larga misura gestito dal Dipartimento della protezione civile e che è ripartito tra le Regioni a seconda del rischio sismico che le riguarda.

e finalmente le università possono veder finanziati i loro progetti sulla valutazione, sulla previsione e sulla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico. Tutto questo, però, evidentemente non era stato previsto nell'organizzazione del fondo nazionale.

più incisiva e perché ci sia stato bisogno di un articolato scritto e pensato rapidamente dalla nostra Commissione e dalla relatrice Di Giorgi. Sono tutti interrogativi che ci poniamo e che vengono in parte

quella perplessità che ho cercato di illustrare in questo breve intervento. Cerchiamo di essere più coerenti nei nostri interventi legislativi. Cerchiamo di sostenere il mondo della ricerca ricerca e di implementare e promuovere davvero la prevenzione, senza attendere sempre, purtroppo, la successiva catastrofe. Cerchiamo di sostenere il mondo accademico e i nostri ricercatori, che sono peraltro giovanissimi e molto richiesti all'estero. Confermo quindi il voto favorevole di Forza Italia su questo provvedimento e ringrazio in modo particolare gli uffici della Commissione e la senatrice Di Giorgi,

il Governo Renzi ha scelto la strada della prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, e idrogeologico, superando la logica della rincorsa delle emergenze, in questo settore particolarmente importante per l'attività sociale ed economica.

anche a causa dell'opera dell'uomo. Sono rilevanti gli investimenti che sono stati fatti in questi anni, a partire dal 2014, dallo sblocco del Patto di stabilità per i Comuni e gli enti locali che intervengono a prevenire con le loro opere i rischi alla sburocratizzazione dei processi che spesso rischiano di bloccare i cantieri, mettendo poi a serio rischio anche quelle zone dove appunto si era intervenuti. Basta ricordare la tragedia di Genova, tra le altre che si sono succedute nel tempo. C'è poi l'investimento cospicuo non è mai abbastanza, ma senz'altro rilevante - sulla sicurezza dell'edilizia scolastica: oltre 4 miliardi di euro destinati alla messa in sicurezza delle nostre scuole. Con questo intervento il Governo fa un ulteriore passo avanti, accogliendo una legge di iniziativa parlamentare che ha iniziato il proprio percorso alla Camera. Ringrazio la relatrice Di Giorgi e tutti i Gruppi che hanno collaborato e che confermeranno, con il proprio voto

del dissesto e del rischio sismico. Lo studio della geologia, infatti, è a rischio estinzione nelle università italiane e ciò è dovuto al blocco del*turnover* e a quei vincoli troppo stretti posti dalla legge n. 240 del 2010, che ha imposto il limite minimo di almeno 40 tra professori e ricercatori del settore scientifico per la costituzione dei dipartimenti universitari. Ma le scienze della Terra sono un'area disciplinare piccola

È proprio la ricerca che nutre la formazione superiore e che permette di trovare soluzioni e metodi sempre più efficaci di prevenzione e di intervento sul nostro territorio. Il disegno che allenta i vincoli numerici della "legge Gelmini" e apre alla costituzione di dipartimenti omogenei per settore disciplinare con la scienza della Terra, serve proprio a non indebolire la conoscenza degli aspetti geologici e a sostenere Senza professionisti in questo campo avremmo nel futuro costi immensi in termini di vite umane e di denaro, per i frequenti disastri naturali che abbiamo visto susseguirsi negli anni. Per rispondere all'intervento del senatore Bocchino, è proprio in una una visione strategica di intervento e non di rincorsa continua delle emergenze che il Partito Democratico dichiara il proprio voto favorevole su questo provvedimento. Un'altra cosa importante da non sottovalutare è l'incentivazione, in un'ottica anche di orientamento dei nostri giovani, a iscriversi ai corsi di laurea grazie a borse di studio, che si aggiungono al diritto allo studio che finalmente, nella prossima legge di stabilità che arriverà in Assemblea, troverà nuovamente risorse importanti

già approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore, senatore Martini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Signor Presidente, farò una breve relazione. Vorrei ribadire che il Senato è riunito oggi per approvare in via definitiva

propone all'Assemblea di votare il testo così com'è uscito dalla Camera, senza ulteriori modifiche, per accelerare e completare l'*iter* di approvazione. Intorno all'oggetto del provvedimento si è sviluppata una discussione costruttiva e collaborativa da parte di tutti i Gruppi, che ha consentito di mettere a fuoco alcuni punti interessanti. Il primo riguarda la figura di Antonio Gramsci, sulla quale non credo sia necessario tornare a lungo, in quanto personaggio che tutte le culture politiche tutti i Gruppi considerano tra le più importanti del Novecento italiano in termini politici e anche resistenziali. Posso solo aggiungere una breve nota sull'attualità del suo pensiero legato al fatto che Gramsci visse in tempi tempestosi e di grandi cambiamenti: subito dopo la fine della Prima guerra mondiale, ci fu la vittoria della rivoluzione bolscevica, la scissione del mondo socialista e l'avvento del fascismo. Tutto era in grande movimento, con un sconvolgimento continuo dello scenario politico e culturale. Anche noi viviamo tempi abbastanza simili, con grandi cambiamenti

Gramsci affrontò questi tempi con la forza del pensiero e con un'attenta analisi dei fenomeni. Il suo pensiero andò e va ancora oggi molto oltre il marxismo e credo sia riconosciuto come pensiero valido da tutte le correnti politiche e culturali del nostro tempo. tempo. È una risorsa utilissima anche ai nostri giorni. È giusta l'esigenza di velocità e prontezza, ma è anche grande il bisogno di pensiero e di profondità.

il prossimo 8 novembre, tra pochi giorni, saranno esattamente novant'anni dall'arresto che Gramsci subì dal regime fascista e sarebbe un modo degno per ricordare la sua battaglia contro la dittatura.

La Commissione ha ritenuto giusto non modificare il testo per renderlo immediatamente vigente impegnando, invece, il Governo (tramite un ordine del giorno), a trovare altri modi e occasioni per riconoscere e valorizzare comunque

Una terza questione ha riguardato la discussione sulla necessità o no di sostegni finanziari a queste iniziative; è prevalsa l'idea di confermare la linea scelta alla Camera di non stanziare fondi in occasione di questo riconoscimento al fine di rimarcare il carattere simbolico e di messaggio culturale di tale scelta, per sottrarre questo riconoscimento a possibili polemiche politiche sull'attribuzione di risorse a questa o altra fondazione e per non ritornare alla Camera e creare imbarazzi, visto che in quella sede era stata chiaramente scelta la via di infine nella nostra discussione una riflessione sulla legislazione relativa alle dichiarazioni di monumenti nazionali. È stata evidenziata - in particolare grazie ad un'iniziativa dei colleghi del Movimento 5 stelle, ma anche di altri colleghi - la necessità di darsi una normativa chiara, non aleatoria e definitiva sul riconoscimento di questi monumenti. il problema si pone e la Commissione ha approvato un ordine del giorno, che il Governo ha fatto proprio, che va nella direzione di aprire una riflessione sul tema e di definire quindi una nuova, complessiva modalità. In conclusione, Presidente, vorrei ringraziare anch'io, come si fa in queste occasioni (ma lo faccio veramente di cuore), tutti i colleghi della Commissione per i contributi che sono stati dati, per il clima positivo che si è instaurato tra di noi, che ha portato alla decisione della Commissione di non modificare il testo. Ringrazio anche il Governo per aver accolto le sollecitazioni volte ad aprire una riflessione su tutta la legislazione relativa ai monumenti nazionali e per aver partecipato attivamente alla nostra discussione. Auspico quindi che si possa oggi con un largo consenso, come già avvenuto alla Camera, concludere l'*iter* di questa legge, che non è sicuramente un grande atto normativo, ma un significativo riconoscimento simbolico in un momento in cui anche i simboli hanno la loro importanza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dovrebbe essere un onore e un privilegio per tutti noi trovarci qui per ricordare e rendere omaggio ad Antonio Gramsci, uno dei più importanti intellettuali italiani del ventesimo Filosofo, storico, giornalista e politico, l'eredità che Gramsci, nel corso della sua breve esistenza, ha lasciato all'Italia è assolutamente impareggiabile. Grazie alle sue grandissime capacità, alla sua profondità di pensiero, all'accuratezza delle sue analisi sociologiche, politiche ed economiche, e alla sua capacità divulgativa, ogni suo scritto, ogni sua idea è ancora oggi fonte di riflessione per tutti noi. L'anno prossimo ricorrerà l'ottantesimo anniversario della sua scomparsa e voglio augurarmi che la decisione di dichiarare la Casa Museo di Antonio Gramsci in Ghilarza, un monumento nazionale, dopo essere stata dichiarata dalla commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna bene di interesse culturale,

Egemonia, società civile, riforma intellettuale e morale, intellettuale organico, blocco storico, nazionalpopolare: tutte queste locuzioni, tutte questi modi di dire vengono da Gramsci e ancora oggi sono di uso comune, seppur non sempre nell'accezione originaria da egli pensata Questo testimonia come il suo pensiero giunga sino ai giorni nostri, fino ad influenzare in maniera determinante il linguaggio di tutte le categorie, giornalisti, politici, storici, filosofi, che Gramsci riassumeva in un'unica persona. Vorrei soffermarmi in particolare sul concetto di egemonia, termine introdotto nel linguaggio comune proprio da Gramsci, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, dove ancora oggi i suoi scritti vengono studiati: basti pensare che la bibliografia internazionale a lui dedicata conta oltre 20.000 pubblicazioni. L'egemonia culturale teorizzata da Gramsci indicava che, attraverso la capacità di orientare la mentalità, l'elaborazione simbolica, gli stili di vita e i linguaggi delle masse, i gruppi dirigenti consolidano e stabilizzano la loro supremazia. allora, fare una riflessione sulla democrazia del presente e del futuro: una democrazia che, purtroppo, deve fare troppo spesso i conti con il populismo, la manipolazione del consenso, la semplificazione dei messaggi, la suddivisione tra buoni e cattivi. Questo scivolamento della democrazia può essere arginato solo attraverso l'educazione delle masse e lo sviluppo di una cultura democratica e popolare di cui Gramsci è stato il primo teorizzatore. Le sue riflessioni sul consenso, sulla necessità di formulare un linguaggio e un progetto politico culturale in grado di tradurre i progetti politici in idee semplici e accessibili anche all'ultimo dei cittadini devono essere la stella polare della politica odierna, così come l'accrescimento della cultura, principale strumento di emancipazione e di libertà. allora, ha ancora oggi molto bisogno di Antonio Gramsci perché egli - come hanno già ricordato i colleghi della Camera dei deputati - è un monumento, ma non è una statua, e il suo non è un pensiero pietrificato nel Novecento, ma un complesso di idee in continuo movimento e di profonda attualità. Dichiarare monumento nazionale la casa di Ghilarza, dove egli visse, a partire dal 1898, gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza, ovvero gran parte della sua breve esistenza, serve a rafforzare la memoria di chi deve ricordare. In questo caso, è la Nazione tutta che deve ricordare un personaggio che l'ha fatta

Antonio Gramsci rientra tra le grandi personalità del Novecento: come Gobetti, Einaudi, Pertini che, pur essendo figure di parte, sono diventate un simbolo per tutti gli italiani. Non vi è quindi alcun bisogno di essere gramsciani, di essere di sinistra per comprendere le ragioni alla base di questo disegno di legge. Non serve condividerne l'ideologia per trovare giusto, e addirittura necessario, approvare questo provvedimento, perché ritengo sia giusto e necessario che una Nazione compiuta celebri e ricordi tutti i suoi grandi uomini. Mi auguro che la politica odierna, certo molto lontana da quella che voleva Gramsci, possa essere promotrice di cultura e memoria condivisa. Concludo questo mio breve intervento augurandomi che quest'Assemblea proceda con lo stesso spirito di condivisione che si è manifestato alla Camera dei deputati. È anche con i simboli, infatti, che si nutre una cultura nazionale condivisa. Per la Repubblica italiana la casa di Ghilarza è importante, perché Antonio Gramsci rappresenta una figura indimenticata e indimenticabile della nostra storia. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione la relazione svolta dal senatore Martini, incaricato di

gli spunti di riflessione, siano tutti condivisibili. Tra l'altro, il senatore Martini ha rimarcato la grande capacità della Commissione di convergere su tematiche condivise, quale, appunto, quella all'ordine del giorno. del carisma, ma anche del valore storico, filosofico e culturale in senso lato della figura e dell'opera di questo grande pensatore del Novecento, possa

appartenente a una determinata corrente politica, può sicuramente essere da noi incentivato per favorirne la memoria. Da questo punto di vista, ritengo che

importanti dal punto di vista della letteratura e del riconoscimento del suo pensiero, contenute nell'opera «Quaderni del carcere». Ci sono tutti i presupposti affinché quella cella possa essere intitolata e quanto meno riconosciuta con un apposito provvedimento istituzionale, quindi formale, affinché se ne preservi la memoria.

sistema complesso, e in alcuni punti controverso, di riconoscimento dei beni monumentali che possono essere elevati alla

vivono ancora gli eredi, i Carrara Verdi, ed è a disposizione dei visitatori tutta la storia di Verdi, la stanza di Giuseppina Strepponi, la sua, tutto il patrimonio musicale, il pianoforte, il famoso busto di Gemito che rappresenta Verdi pensoso, il letto di morte, gli autografi del Manzoni e il carteggio tra Manzoni e Verdi. Credo che se c'è un luogo che merita di diventare monumento nazionale sia quella

è conservata tutta la documentazione, la storia, perfino il mobilio originale d'epoca acquistato da lui oltre a tutti i suoi scritti agrari, e ricordo che era un grande imprenditore, un grande innovatore anche dal punto di vista dei fondi che gestiva personalmente.

È iscritto a parlare il senatore Uras,

Peraltro, della casa natale è rimasto un muro originario e vi è stato realizzato un centro, sostenuto con finanziamenti della Regione sarda, di discussione, dibattito culturale e di memoria dello stesso Gramsci.

del pensiero di Antonio Gramsci, oltre alla sua attualità. Voglio però fare una riflessione su questa personalità: è un giovane povero di un Paese poverissimo e periferico di una regione periferica come la Sardegna. serie di vicende negative relative alla sua famiglia. Il padre è colpito da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Le condizioni di povertà della sua famiglia sono di una precarietà assoluta. Nonostante questo, avvalendosi di pochissimi aiuti, Antonio Gramsci studia, in una difficoltà che diventa anche difficoltà fisica nell'affrontare gli studi. Il Il suo corpo è lacerato da malattie, che ne condizionano la capacità produttiva e, nonostante tutto, studia, si diploma al Liceo classico Dettori di Cagliari e si iscrive all'università di Torino, dove partecipa ai moti

in una condizione disperata, scarcerato perché alla vigilia della morte. È quindi morte. È quindi impressionante la qualità e la capacità di pensiero e di elaborazione, anche letteraria,

pezzettini di matita, su quaderni che gli vengono consegnati dal direttore del carcere, in una condizione assolutamente fuori dal comune. Eppure egli è uno degli autori italiani più tradotti al mondo, condividendo questo primato, Niccolò Machiavelli. Questo è Gramsci. Se non si capisce che dalle situazioni di maggiore difficoltà possono nascere spiriti, personalità culturali intellettuali di questo spessore, non si capisce neppure la realtà dei nostri giorni. Quando vediamo le moltitudini dei disperati, poniamoci il problema che forse, tra quelle moltitudini, ci sono tanti Gramsci, ovvero tanti giovani in grado di dare un contributo intellettuale nella storia del mondo, come ha fatto Gramsci. il provvedimento in esame, costituito da un solo articolo, dichiara monumento nazionale la Casa Museo di Gramsci sita

e, come centro di documentazione, ha dato impulso anche alle ricerche sulla sua vita e sul suo pensiero, facendo così conoscere la storia del movimento operaio italiano e internazionale. Oggi, a fruire di questo bene di inestimabile valore sono soprattutto gli studenti, che in questo modo possono scoprire il valore che la figura di Antonio Gramsci ha avuto, sia dal punto di vista del pensiero politico, sia come giornalista impegnato nell'edizione piemontese dell'«Avanti» ed in seguito dell'«Ordine Nuovo», che divenne «il giornale dei Consigli di fabbrica». Nei suoi articoli gli operai ritrovavano «la parte migliore di se stessi», perché contenevano e trasmettevano sentimenti, volontà, passioni reali di chi voleva diventare libero. Nel presente disegno di legge si intende dichiarare monumento nazionale la Casa Museo di Gramsci. Questa posizione è condivisibile, ma risulta esserci un vuoto normativo. L'istituzione dei primi monumenti nazionali risale addirittura alla legge n. 3096 del 7

Inoltre le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento a beni qualificati come monumenti nazionali: in particolare, la legge n. 1089 del 1939 introduceva la nuova nozione di interesse storico-relazionale, sulla quale anche il Ministero dei beni e delle attività culturali ha espresso le proprie perplessità nel parere del 6 marzo 2006. È pertanto necessario procedere 6 marzo 2006. È pertanto necessario procedere alla definizione di una legislazione nazionale, che istituisca un quadro normativo di riferimento e una precisa definizione di monumento nazionale, superando l'attuale incongruenza normativa, idonea solo a garantire il riconoscimento di mere onorificenze, nonché a produrre provvedimenti circoscritti come questo in esame. Quando si parla di patrimonio culturale, quindi, il quadro normativo presenta quasi sempre delle lacune che inficiano la piena e coordinata fruibilità dei beni culturali. Per tutta risposta neanche la riforma costituzionale Boschi-Renzi-Verdini (contrariamente a quanto viene sbandierato negli *spot* e negli interventi televisivi dai membri del Governo) risolve il problema, nella revisione del Titolo V, sulla quale andremo a votare il prossimo 4 dicembre, la valorizzazione del patrimonio culturale è una materia che viene assegnata in capo allo Stato, mentre la sua promozione viene assegnata agli enti locali. Questa impostazione produrrà innumerevoli conflitti di competenza davanti alla Corte costituzionale, che sarà impegnata a dirimere il sottile e difficilissimo confine tra «promozione» e «valorizzazione». Ritornando alla definizione di «monumento nazionale» apprezziamo che il Governo abbia riconosciuto l'importanza di una legislazione nazionale e abbia accolto in 7a Commissione un ordine del giorno

degli immobili dichiarati monumenti nazionali secondo la normativa vigente» (articolo 54, comma 1, C'è da considerare inoltre l'appartenenza della Casa Museo al patrimonio immobiliare della Fondazione Berlinguer, che è strettamente legata ad una storia e ad una tradizione politica

con questo disegno di legge, la Fondazione potrebbe accedere in modo privilegiato ai fondi pubblici. Pertanto, auspichiamo che il Governo predisponga rapidamente, in ottemperanza all'ordine del giorno accolto, tali norme, istituendo un quadro normativo di riferimento e fornendo fornendo una precisa definizione di monumento nazionale, al fine di evitare iniziative legislative circoscritte come quella in esame che, seppur lodevoli dal punto di vista storico-culturale, potrebbero essere mosse anche da ben altri interessi, nonché garantire l'inalienabilità dei monumenti nazionali e la necessaria trasparenza delle risorse finanziarie che vengono ad essi destinate. iscritto a parlare il senatore Lai. è nell'indifferenza che sono nati e si sono consumati i fatti più tragici della nostra storia. Non è certo un caso che Antonio Gramsci, con le parole chiare e forti di chi ha vissuto in prima persona il drammatico della dittatura nazifascista, ha voluto significare il suo odio verso gli indifferenti, perché, come scrisse Gramsci, «l'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita». E forse oggi avrebbe aggiunto che è conformismo. Quel monito, quella sua distanza ostile verso gli indifferenti, resta un lucido insegnamento anche per la fase storica che viviamo, nella quale proviamo a combattere il distacco e la disaffezione, consapevoli anche del ruolo e delle responsabilità della politica, ma coscienti che solo dalla buona politica, dalla politica che consente la partecipazione, che spinge alla responsabilità e che stimola la passione, può arrivare il contrasto all'indifferenza, che oggi confina con la rassegnazione; coscienti che la politica ha un indifferibile bisogno di rafforzarsi in quelle fondamenta valoriali, di libertà e di democrazia, che sono la premessa per mantenere coesa la comunità nazionale e forse, oggi, quella europea. Questo è certamente un cuore pulsante del pensiero e dell'insegnamento di Gramsci. Per questo, pur nella consapevolezza della diversità di opinioni che si possono manifestare sul pensiero di Antonio Gramsci, ritengo che sarebbe riduttivo affrancare solo come simbolico il provvedimento sul quale siamo stati chiamati a esprimerci. Per noi sardi Gramsci è prima di tutto un sardo, parte del nostro orgoglioso essere e sentirci popolo. Ma sappiamo che Gramsci è un intellettuale nazionale, ne siamo consapevoli. Il suo pensiero e la sua opera rappresentano un patrimonio inestimabile per la nostra storia, la nostra cultura e il nostro vivere in un Paese che ha molto ben chiari i valori della democrazia, della libertà e dell'antifascismo e non li vuole dimenticare. Gramsci è parte della cultura nazionale e parte fondante di un pensiero che si è diffuso oltre i confini nazionali. Come ha ricordato un collega, Gramsci è uno degli autori italiani più tradotti nel mondo. Gramsci è soprattutto un punto di riferimento per chi vuole dare valore all'idea che si possa aiutare la formazione della coscienza civica di ogni singolo cittadino. Il suo pensiero rende chiara l'idea del significato più puro e concreto del concetto di militanza politica, ma anche del vivere, da cittadino semplice, al servizio del proprio Paese e della comunità, anche nel nostro tempo. Oggi, dunque, discutiamo sulla proposta di dichiarare monumento nazionale la casa nella quale è nato e vissuto. Quella casa è già un simbolo, sicuramente per tutti i sardi ma anche per tutti gli italiani che vogliono vivere e respirare i luoghi in cui lui si è formato. Quella di oggi è un'occasione per riconoscere a quel luogo l'importanza che merita Gramsci anche per il Parlamento, vale a dire per ciò che rappresenta la nostra istituzione e per ciò che ha rappresentato Gramsci come deputato. Come è stato ricordato, l'8 novembre sarà il 90° anniversario dell'arresto di Antonio Gramsci da parte del regime fascista. È una data che deve far parte della nostra storia e dobbiamo compiere ogni sforzo possibile perché rimanga sempre viva. Ci ricorda un atto che ha colpito non solo l'uomo in sé, ma anche l'istituzione che rappresentava: quello stesso Parlamento che oggi può restituire una parte della dignità violentata, con la privazione della libertà, al deputato Gramsci.

ma lo si può capire anche entrando in contatto con quell'abitazione, con i luoghi, gli oggetti e la documentazione, che non solo si può visionare, ma è a disposizione di chiunque voglia conoscere bene, profondamente, il pensiero di Gramsci. Con il provvedimento che oggi esaminiamo possiamo dare a tutto questo un significato ancora più profondo, riconoscendo la memoria dei luoghi come spazio ideale dal quale trarre insegnamento per il nostro vivere in un Paese democratico e libero. Lo dobbiamo a quello che ancora oggi Gramsci rappresenta e per quello che può rappresentare in futuro, anche grazie al fatto che quella casa può diventare, con il nostro voto, monumento nazionale. Se questo contribuirà anche solo in minima parte a tenere sempre vivo e accessibile a tutti quello che Gramsci ci ha lasciato in eredità vorrà dire che avremo compiuto un atto che sarebbe riduttivo definire simbolico. Finite le ideologie del Novecento resta nel pensiero, nella sua storia, nel suo esempio, nella sua vita, un insegnamento sulla libertà e sulla democrazia che merita di arrivare integro alle generazioni più giovani.

Signor Presidente, non voglio ripetere quanto è già stato detto molto bene dal relatore e dai colleghi che mi hanno preceduto sull'importanza storica, intellettuale, politica e letteraria di Antonio Gramsci e sull'alto valore simbolico che ha questo riconoscimento. Vorrei solo riprendere un pensiero che è stato, anche questo, molto ben esposto dal senatore Lai nell'ultimo intervento: un Paese che non ha una memoria storica è un Paese facilmente esposto a qualunque genere di estremismo, qualunque genere di estremismo che non può che vedere qualunque cittadino democratico opporvisi. E un modo per fare un'opposizione reale, un'opposizione reale, che si radichi anche nelle future generazioni, è quello di mantenere viva questa memoria storica. Ecco quindi che il provvedimento che oggi viene portato all'esame del Senato assume un significato, particolarmente nei tempi che stiamo vivendo, profondo, ampio ed anche necessario. Vorrei altresì raccogliere due sollecitazioni arrivate dal senatore Liuzzi e dalla senatrice Blundo riguardo alla necessità che ci si doti di strumenti per poter decidere quali beni rientrino tra i monumenti nazionali: quali siano i criteri, in che modo si debba procedere. Non userei il termine «trasparenza», senatrice Blundo, perché credo che nella decisione che oggi il Senato si appresta a prendere non ci sia alcunché di non trasparente se non il riconoscimento di una grande e importante figura della nostra storia. Ma è giusto pensare che il nostro Ministero, anche con l'aiuto e il sostegno delle Commissioni parlamentari, presto si attivi per cercare di definire quali siano questi criteri, criteri, per facilitare non solo il nostro lavoro nel futuro, ma anche il lavoro del Parlamento quando viene chiamato a decidere sulla definizione di monumento nazionale.

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2342 , recante «Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo di Gramsci in Ghilarza»; premesso che il riconoscimento di monumento nazionale di un sito assume valore testimoniale e di esperienza mnemonica; attesa attesa la valenza culturale, storica, politica, letteraria dell'opera "Quaderni del carcere", elaborata da Antonio Gramsci negli anni 1928-1933

proprio per il riconoscimento del valore e della figura di Antonio Gramsci, il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo ordine del giorno. Vorrei ricordare che la figura di Gramsci è apprezzata anche da parti politiche molto distanti dalla sua, come ho avuto modo di appurare, avendo

Non mi resta che appellarmi alla seconda carica dello Stato affinché chiarisca istituzionalmente questa situazione. Non possiamo vivere in un Paese in cui viene detta questa cosa su uno dei giornali a diffusione nazionale *(Commenti dal Gruppo PD)* e si Dopo che il sì al *referendum* è stato favorito già da RAI, Mediaset*,* Sky, da Obama, dall'Unione europea*,* da Goldman Sachs, dalla finanza e dal presidente emerito Napolitano (che ogni volta che apre bocca viene riportato su tutte le prime pagine), trovo inaudito che vi sia il

Grazie, senatore Airola, ringrazio per il suo intervento.

È una prassi di cui il Parlamento non aveva mai sentito l'esigenza ed è stata - io ritengo - istituita per

sono in totale contraddizione con interventi della volgarità che ha contraddistinto l'intervento che ho appena ascoltato di un senatore del

livello. Devo dire che, se pensa veramente di fare un servizio alle istituzioni con queste volgarità nell'Aula del Parlamento... Il Gruppo Partito Democratico, che in questo Parlamento ha la maggioranza relativa, non è mai intervenuto con questi schiamazzi, anche quando da quei banchi vengono a noi insulti gravissimi e ingiustificati*. (Applausi che il Partito Democratico non possa parlare in Aula perché viene interrotto continuamente da persone che stanno in Parlamento senza meritare di esserci *(Applausi dal Gruppo

Detto questo, tutti coloro che sono in questa Assemblea meritano di esserci, perché qualcuno ha votato perché ci fossero: di questo la Presidenza non può che prendere atto.

Non si può neanche dire che i colleghi del Partito Democratico non possono svolgere i loro interventi. Tutti noi che presiediamo i lavori sappiamo che gli interventi si svolgono tutti, anche se a volte in condizioni più